Comunico che, in data 16 maggio 2008, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri:* «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» Onorevoli colleghi, con lettera del 15 maggio scorso, il Presidente della Repubblica ha trasmesso alla Presidenza del Senato una petizione a lui inviata, sottoscritta da più di un milione di cittadini, volta a chiedere il riconoscimento alle famiglie di agevolazioni, anche di natura economica e fiscale, al fine di favorire il formarsi di nuovi nuclei familiari e l'adempimento dei relativi compiti. Nella sua lettera, il Presidente della Repubblica sottolinea inoltre la necessità che il nuovo Parlamento affronti i temi delle politiche della famiglia, con particolare attenzione ai problemi dell'occupazione femminile, della indispensabile coesistenza tra vita familiare e vita lavorativa, nonché della complessiva crescita del sistema nazionale dei servizi socio-educativi per l'infanzia, confidando che, in sede di programmazione dei lavori parlamentari, possa essere assicurato un esame tempestivo delle iniziative legislative che saranno presentate in materia. Nella convinzione che il Senato della Repubblica nella XVI legislatura riserverà un'attenzione particolare a questo tema di straordinario interesse e attualità, ho assicurato al Presidente della Repubblica che la petizione medesima sarà immediatamente trasmessa alle competenti Commissioni, non appena costituite. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 5 giugno. Questa mattina inizierà l'esame del decreto-legge sul trasporto aereo, con eventuale prosieguo nella odierna seduta pomeridiana e, se necessario, domani mattina non oltre le ore 11,45. La prossima settimana, nella seduta antimeridiana di martedì 27 maggio, appositamente convocata alle ore 11, il Ministro degli affari esteri renderà una informativa al Senato sui recenti sviluppi della situazione in Libano. Potranno successivamente intervenire i Gruppi per dieci minuti ciascuno. Dal pomeriggio di martedì 27 maggio e nelle successive sedute di mercoledì 28 e giovedì 29 maggio, saranno discussi i decreti-legge, attualmente all'ordine del giorno della Camera dei deputati, ove approvati e trasmessi in tempo utile, in materia di segretezza del voto nelle consultazioni elettorali, trasporti ferroviari regionali, protezione civile e attuazione degli obblighi comunitari. Ove non conclusi nel corso della prossima settimana, tali decreti proseguiranno la settimana successiva, nelle sedute previste per mercoledì 4 e giovedì 5 giugno. Per quanto riguarda il sindacato ispettivo, nelle sedute pomeridiane di giovedì 29 maggio e giovedì 5 giugno saranno svolte rispettivamente interpellanze e interrogazioni e interrogazioni a risposta immediata. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Regolamento, le Commissioni permanenti sono convocate, per la loro costituzione, nella giornata di domani, giovedì 22 maggio, nei seguenti orari:

Comunico inoltre che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è convocato per la sua costituzione, presso palazzo San Macuto, domani alle ore 14,30.

Presidente, colleghi, concordo con l'intervento del senatore Zanda:

Zanda, reiterando peraltro - come sa - una segnalazione che mi ero permesso di fare riservatamente, anche a seguito della decisione presa dalla Camera dei deputati di dedicare ad Aldo Moro, in forma solenne,

Collega Zanda, colleghi senatori, la Presidenza del Senato, ovviamente a nome del Senato, ha preso parte a momenti commemorativi della vicenda relativa all'eccidio del grande Aldo Moro. In ogni caso, sono prontissimo a consultare i colleghi Capigruppo per individuare tutti assieme un momento commemorativo dello statista al fine di giungere, in tempi brevissimi e all'unanimità, ad un percorso che possa impegnare l'Aula. Tra l'altro, l'iniziativa mi vede pienamente partecipe e in piena sintonia con la richiesta del senatore Zanda. Pertanto mi riservo, in maniera probabilmente informale, anziché convocare una Conferenza dei Capigruppo, di ascoltare i colleghi per individuare in maniera ufficiosa un un percorso, una iniziativa che impegni l'Aula al più presto, compatibilmente con i lavori parlamentari. Ritengo sia nostro dovere, ed è dovere di quest'Aula, trovare gli spazi e i tempi per questo importante momento.

il decreto-legge al nostro esame consente alla società Alitalia di utilizzare un prestito ponte di 300 milioni di euro per far fronte alle necessità derivanti dall'onere di continuare a svolgere un servizio pubblico fondamentale. L'intervento è parimenti finalizzato a non compromettere la conclusione del processo di privatizzazione della società Alitalia, privatizzazione che il Governo appena insediato ha dichiarato di voler perseguire. Sono note al mercato le condizioni economico-finanziarie della nostra compagnia di bandiera. La criticità della situazione risulta aggravata, rispetto alle più recenti previsioni, da fattori economici esterni, in particolare dal fortissimo aumento del prezzo del carburante, che ha sensibilmente impattato sulle prospettive di riduzione delle perdite operative e sul mantenimento della liquidità ritenuta necessaria. Il prestito di cui si parla ha caratteristiche di mercato, non comporta - a mio parere questo è molto importante sottolinearlo - né effetti sui saldi di finanza pubblica, né variazioni di bilancio. Il prestito - com'è evidenziato nella relazione tecnica - dovrà essere rimborsato entro il corrente esercizio (quindi entro il 31 dicembre 2008), maggiorato di un tasso di interesse nella misura prevista dalla specifica disciplina comunitaria richiamata nel decreto-legge in questione. Il dibattito svolto in Commissione, onorevoli colleghi, è stato volutamente circoscritto ai contenuti del provvedimento, ancorché sia ben presente a tutti i colleghi che hanno partecipato ai lavori della Commissione l'esigenza di affrontare al più presto le questioni di merito, di sistema, cioè le questioni politiche legate al futuro e alle prospettive della società Alitalia. Non appena le Commissioni permanenti saranno insediate, ritengo che questo argomento sarà tra i temi centrali del dibattito politico. In questo senso, il Governo, sollecitato a dare risposta ai tanti quesiti legati al processo di privatizzazione, al piano industriale di cui da tempo si parla, all'ingresso di nuovi partner finanziari e gestionali, ha confermato l'impegno a riferire al più presto in Parlamento sullo stato dell'opera. Con l'intesa, quindi, di tornare al più presto a confrontarci su un tema che ha occupato tanto spazio nella recente campagna elettorale e che riveste una straordinaria importanza in un settore strategico per lo sviluppo del nostro Paese, ci occupiamo quest'oggi del decreto-legge n. 80, che si prefigge di garantire - come ho già detto - la continuità di un servizio pubblico essenziale in presenza di fattori esterni che hanno sensibilmente peggiorato l'equilibrio di gestione della nostra compagnia di bandiera. Il consenso unanime che con grande soddisfazione abbiamo registrato in Commissione sul testo proposto dal Governo non ha impedito alla Commissione stessa di approfondire questioni che, sollevate da vari colleghi, hanno ricevuto già in quella sede - e credo sarà reiterata in Aula - una puntuale e precisa risposta da parte del rappresentante del Governo. Mi riferisco, in particolare, all'interesse che la Commissione ha rappresentato di avere da parte del Governo assicurazioni che l'intervento proposto non corra il rischio di essere giudicato una forma di aiuto di Stato dalla Commissione europea. Ancora, altri colleghi, sempre nel dibattito svolto in Commissione, nel rimarcare la necessità di un intervento organico ed urgente, hanno evidenziato con preoccupazione il peggioramento dei conti di Alitalia secondo l'evidenza emersa nell'ultimo Consiglio di amministrazione della società dalla lettura dei dati della relazione trimestrale e, conseguentemente, hanno lamentato il fatto che il Governo non fosse già oggi in condizione di chiarire le sue scelte, cioè le intenzioni che si hanno nel perseguire il rilancio della società in questione. In sede di replica, tuttavia, il rappresentante del Governo ha confermato già in Commissione di aver avviato un proficuo confronto con la Commissione europea e di aver difeso in quella sede la tesi che l'intervento non può configurarsi come aiuto di Stato, ma piuttosto come un legittimo intervento finanziario a scadenza, finalizzato solo e soltanto a superare la fase acuta di crisi nella prospettiva di realizzare a breve un nuovo piano industriale. Va in questa direzione l'insieme di osservazioni teso a rimarcare l'esistenza di problemi riconducibili alla difesa della coesione territoriale, alle esigenze territoriali più in generale, ai pericoli di gravi turbamenti sociali, alla necessità di garantire al nuovo Governo, signor Presidente, dopo una stasi dovuta alla

anche se, per ragioni tecniche, fu approvato il 23 aprile scorso dal Governo precedente. Signor relatore, colleghi, ricordo molto bene il 23 aprile; ricordo non solo i dettagli con cui si è arrivati a questa decisione, ma anche l'imposizione della cifra, che ci è stata richiesta dai vincitori delle elezioni che si apprestavano ad assumere le redini dell'Esecutivo,

che l'erogazione di 300 milioni di euro è stata data «per non comprometterne la continuità operativa nelle more dell'insediamento del nuovo Governo» ponendo quest'ultimo «in condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società». società». Cari colleghi, un finanziamento ponte, come dice la parola, presuppone che ci sia un'altra sponda e l'altra sponda che avevamo individuato era quella della vendita, dopo la gara andata deserta, e della trattativa con Air France. Oggi, grazie anche al fatto che il tema Alitalia è stato usato in tutta la campagna elettorale, in nome di un'italianità che non si capisce bene cosa sia, è stata fatta fallire, esattamente per le prese di posizione reiterate del Presidente del Consiglio, giudicando la proposta avanzata spesso in alleanza anche con le varie sigle sindacali, che nulla si sono fatte mancare per far fallire la trattativa stessa. Oggi quindi non c'è niente sul tavolo. Per questo non è un prestito ponte, perché manca l'altra sponda. A distanza di un mese dal 23 aprile, nulla appare di strabilianti e mirabolanti cordate italiane, ammesso che una cordata italiana abbia non solo i fondi per comprare Alitalia ma soprattutto gli investimenti necessari per reimmettere il nostro Paese nel traffico aereo globale, perché di questo parliamo, non di farne una minicompagnia regionale.

di inserire il nostro Paese e l'Alitalia in questo *network* di traffico aereo globale - perché questa è la sfida - oggi non è più sul tavolo;

È semplice: Alitalia, da anni, distrugge, non crea valore aggiunto. In sette degli ultimi otto esercizi, contando anche il 2007, ha registrato perdite, solo perdite. Alitalia ha dunque perduto il connotato costitutivo dell'impresa; in senso tecnico, dovremmo definirla come un'azienda di consumo, al pari di una famiglia o di un'opera benefica, pagata dalla generosità degli italiani per imposizione di leggi. Non solo, ad aggravare un quadro già a tinte fosche, oggi gli analisti internazionali ci avvertono che ogni giorno che passa il valore del *brand* Alitalia si assottiglia, ogni mese perde potere di contrattazione. un'analisi convalidata anche dagli ultimi dati, che indicano che la compagnia ha chiuso il primo trimestre dell'anno con una perdita di 215 milioni di euro, dovuta in parte al rincaro del carburante. È vero, senatore, però il rincaro del carburante colpisce tutte le compagnie del mondo, è di tutta evidenza, ed è per questo che tutte le compagnie del mondo vedono il loro margine assottigliarsi ed ogni giorno che passa sarà più difficile trovare acquirenti adeguati al traffico aereo da gestire, non adeguati a metterci solo qualche soldo. C'è anche un'ulteriore svalutazione di 97 milioni di euro del valore della flotta. Se a questo si aggiunge che oggi il valore di mercato dell'Alitalia è di appena 800 milioni mi sembra che il quadro diventi nero per i contribuenti italiani, per gli imprenditori (che hanno bisogno di connessioni), per i cittadini italiani e per i turisti che eventualmente volessero venire nel nostro Paese. Credo si sia trattato di una pagina di irresponsabilità da parte vostra. Voi conoscete molto bene la situazione dell'Alitalia; intanto l'avete governata per cinque anni, dal 2001 al 2006, 2006, proponendo piani di ristrutturazione falliti ed ottenendo, peraltro per l'ultima volta, una congrua iniezione di aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea, che all'epoca, nel 2005, La prossima scadenza può essere eventualmente il 2011. Colleghi, è su questo aspetto che mi soffermerò di più. Intanto non è un prestito ponte e, al di là del vocabolario, la relazione indica chiaramente che cosa

La Commissione europea ha espresso già tutte le sue perplessità sulla congruità dell'operazione e aspetta, entro il 30 maggio, non solo la notifica formale ma una serie di spiegazioni che vanno fornite per evitare l'adozione di una ingiunzione di recupero a titolo provvisorio ma a carattere vincolante, come sapete, colleghi, vista anche la reazione di Ryanair e non solo, perché si aspetta anche quella della SAS. la possibilità di adire direttamente alla Corte di giustizia quindi mi auguro, ci si augura, ci auguriamo tutti che questo ponte finalmente appaia, ma entro il 30 maggio perché altrimenti credo che scadranno i tempi.

che hanno segnato tutta la campagna elettorale. Ma che vorrà mai dire italianità? Forse vuol dire proprietà? Per me italianità vuol dire servizio agli italiani, vuol dire che gli italiani devono potersi muovere e devono poter volare non ai prezzi attuali e con un servizio come quello dell'Alitalia. Questa è l'italianità che ci interessa. L'italianità dei consumatori e dei cittadini italiani, indipendentemente dalla nazionalità del passaporto delle strabilianti cordate italiane, o magari russe, che non si sono mai verificate.

non parteciperà perché altro avevamo individuato, altro avevamo ottenuto. Voi l'avete fatto saltare, voi dovete risolvere oggi questa situazione per i cittadini e per i consumatori italiani.

Il Governo, nella Commissione speciale, ha fornito ampie garanzie su questo; ritengo che un nuovo Governo che si insedia debba avere anche del tempo materiale per poter proporre le varie questioni. voglio aggiungere che il tema trattato è importantissimo, in modo particolare per noi della Lega che abbiamo rivendicato un ruolo fondamentale per l'aeroporto di Malpensa,

conto: si tratta di 300 milioni di euro. Non si parla di pilastri, come ricordava qualcuno in Commissione, o di sponde mancate, come ha detto lei. Si tratta di

Stamattina rischiamo di ripetere tutti le stesse cose, però abbiamo visto che, essendo in presenza della gravissima situazione economico-finanziaria di Alitalia, bisogna far fronte, nell'immediato, al fabbisogno di liquidità.

non si doveva verificare. In secondo luogo, bisogna garantire la continuità di un servizio, quello del trasporto pubblico, anche se è riservato, sempre e comunque, ad una ristretta fetta di società:

dovrebbe contribuire alla conclusione del processo di privatizzazione di Alitalia. Lo Stato, quindi, concede ad Alitalia un prestito a breve termine che deve essere restituito. Noi ci auguriamo e crediamo fortemente che questi soldi vengano restituiti entro la fine dell'anno, guai se non fosse così! La compagnia di bandiera (che ha ricevuto aiuti di Stato

non dovrà avere effetti negativi sulla finanza pubblica.

di fronte al rischio di un fallimento. Quindi, per noi si tratta di una ulteriore opportunità concessa alla compagnia di bandiera, propedeutica ad un rilancio anticipato dell'azienda che salvaguardi il ruolo - per noi importante - dell'aeroporto di Malpensa. Alitalia dovrebbe tornare a fornire servizi di trasporto efficienti ed economicamente validi, in una condizione sul territorio rispetto a tutti gli altri attori del settore, tenendo presente che il mercato del trasporto aereo in Italia è potenzialmente molto redditizio; non si devono più commettere gli errori del passato, quando una gestione esclusivamente clientelare e di spartizione partitocratica dell'intero settore ha determinato conseguenze fallimentari e disastrose. Pertanto, approvato questo provvedimento, la partita tornerà - anzi è già - nelle mani del Governo per la privatizzazione. Il Ministro dell'economia intende affrontare la crisi con una soluzione fondamentalmente italiana e privata;

tenga presente che l'obiettivo di Air France era quello di affossare Malpensa, con il trasferimento dei voli su Fiumicino ed il conseguente incremento dei voli dell'aeroporto di Parigi.

del Veneto, che sono una ricchezza per il Paese intero, dovranno ricevere la giusta attenzione da parte del nuovo Esecutivo. I posti di lavoro a rischio sono circa 6.000, molti di più se si considera l'intera area vasta di Milano, Novara e Varese e l'occupazione indotta dalla presenza di quello che è il più importante aeroporto dell'Europa centro‑meridionale. Desidero inoltre evidenziare che da

tutte le componenti istituzionali, economiche e sociali hanno fatto sentire la propria voce per rafforzare le dotazioni infrastrutturali al fine di favorire la proiezione internazionale del territorio. La realizzazione di Malpensa 2000 ha significato a suo tempo la creazione di uno scalo in grado di competere con gli altri aeroporti europei. I dati che ci vengono forniti su Malpensa sono del tutto positivi e in crescita.

la Lega Nord Padania ha sempre assunto una posizione critica nei confronti di Alitalia. Rivendico al nostro movimento politico di aver

onorevoli colleghi, il consenso unanime sul contenuto del decreto che ci ha illustrato il relatore, il collega Grillo, non ci ha impedito in Commissione di esporre le nostre gravi preoccupazioni sulla situazione che si è venuta a determinare. Abbiamo inutilmente chiesto l'audizione del Ministro dell'economia e del presidente di Alitalia in Commissione: era stata fissata per la giornata di ieri, ma è stata poi disdetta con la promessa generica di compiere lo stesso atto davanti alla Commissione di merito nei prossimi giorni. La nostra non era un'istanza dilatoria, giacché abbiamo motivato il nostro voto favorevole dal punto di vista tecnico per la necessità che si è venuta a determinare per le ragioni che conosciamo, ma un'istanza fondata su preoccupazioni serie. Vi era e vi è la necessità inderogabile di chiarire che cosa il Governo vuole su questa importante questione. Le posizioni espresse durante la competizione elettorale ci sono note e la situazione della compagnia nella sua gravità ci è altrettanto nota. Ad oggi, signor Presidente, il capitale di Alitalia

emerso che il capitale netto residuo della compagnia ammonta a 96 milioni di euro; considerato che dal 31 marzo ad oggi sono passati 50 giorni, è altamente probabile che il capitale di Alitalia

Aveva ragione l'ex Ministro dell'economia allorquando, nel sollecitare una chiusura rapida di quella vicenda, avvertiva che il tempo che il tempo stava per scadere. Aveva ragione anche quando, nell'ultima audizione che egli sostenne davanti alle Commissioni di merito durante la campagna elettorale, disse che non vi erano le condizioni per concedere questo prestito ponte, anche se poi è stato concesso per evitare il peggio e per aderire alla richiesta pressante che veniva da chi aveva vinto le elezioni e si accingeva ad assumere la carica di capo del Governo. La struttura del decreto formalmente ci dice che vi sarebbero le condizioni per concedere questo prestito sulla base del diritto comunitario, i cui princìpi ci sono noti, ma appunto, per le cose che sosteneva la collega Bonino poco fa, i presupposti sono gravemente minati dal fatto che, ad oggi, non vi è una soluzione: nella sostanza, tutto il supporto motivazionale del decreto richiede la condizione inderogabile che questa privatizzazione si concluda nel giro di pochissimo tempo: la cessione, con conseguente approvazione di un piano industriale, di un piano finanziario di risanamento entro pochissimo tempo. Non è un caso che il il decreto stesso preveda, appunto come *dies a quo* per la restituzione del prestito, il completamento della privatizzazione della società. Il nesso tra il prestito e la necessità inderogabile di concludere questo processo è rafforzato dall'obbligo fissato al comma 3 dell'articolo 1 del decreto, il quale sostanzialmente prevede che tutti i pagamenti pagamenti e le garanzie posti in essere dopo l'entrata in vigore del decreto sono esclusi dalla revocatoria fallimentare, a tutela dei creditori e dei fornitori di servizi della società stessa. Ma perché tale norma operi - questo lo dice la legge fallimentare - occorre che tali atti siano posti in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa o ad assicurare il riequilibrio, per esempio attraverso la cessione del pacchetto azionario, e che la ragionevolezza di tale piano sia attestata da un professionista abilitato. Avremmo voluto sapere e vogliamo sapere dal Governo se il piano previsto dalla legge è stato redatto ad oggi mentre ci accingiamo a convertire il decreto, e quale professionista, sempre ad oggi, potrà attestare la ragionevolezza del completamento dell'*iter* entro tempi strettissimi, per fare in modo che questa norma posta a salvaguardia appunto della società e dei suoi fornitori possa essere interamente operativa. Il Parlamento deve essere garante di questa situazione, controllore anche della trasparenza dell'operazione di cessione, se essa si riavvierà e si concluderà qualora nei prossimi giorni si manifestasse

Ad esempio, in campagna elettorale, alla famosa cordata è stato subito accostato il nome del dottor Ermolli, il superconsulente dalla famiglia Berlusconi e di altre operazioni societarie. Giorni fa il dottor Ermolli ha richiesto documenti contabili ad Alitalia, qualificandosi come incaricato del Presidente del Consiglio. L'istanza è stata rigettata dal consiglio di amministrazione, non essendovi alcuna proposta, non essendo egli latore di una proposta concreta e non essendovi un mandato né da parte di acquirenti, né da parte del Presidente del Consiglio. Ricordo all'Assemblea

di Mediolanum, nonché di presidente di Medusa Film, tutte società riconducibili alla persona del Presidente del Consiglio. Dunque, a che titolo il dottor Ermolli agisce? Ce lo dovete dire. Il Governo ce lo deve dire. Se egli è un consulente privato che agisce per conto di imprese private, vi sarebbero gravi ragioni di opportunità ma, insomma, egli sarebbe libero di agire come ritiene. Se, invece, in base a agisce per conto del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, sono evidenti i gravi e seri problemi; è bene che il Governo ci chiarisca

dell'azienda Telecom. Ecco perché ogni giorno che passa, signor Presidente, si accumulano gravissime preoccupazioni e molti interrogativi. Noi assumeremo iniziative perché è doveroso che il mercato, il Parlamento, il Paese sappiano come stanno le cose

finestra") *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo decreto di 300 milioni di euro che il passato Governo è stato costretto a varare per dare respiro breve ad Alitalia abbiamo infilato in un buco nero miliardi di soldi pubblici, dei cittadini che pagano le tasse. La cordata italiana, annunciata durante la campagna elettorale, ancora non si è materializzata, ma nel frattempo il titolo Alitalia ha subito pesanti oscillazioni di Borsa, tali da configurare ipotesi di *insider trading*, aggiotaggio, turbativa dei mercati. L'ipotesi di una cordata capeggiata da Air One rischia di provocare un danno alla concorrenza ed ulteriori oneri ai consumatori. Voglio solo ricordare che qualora Alitalia venisse aggiudicata alla alla compagnia di volo italiana verrebbe rafforzato il monopolio sulla ricca rotta Roma-Milano, sulla quale un biglietto costa più di un volo Roma-New York.

con i 300 milioni si sale a 4,6 miliardi di euro infilati in un colabrodo e chissà se saranno mai restituiti. Se l'Europa non blocca il prestito ponte perché viola le norme sulla concorrenza, l'italianità, per chi ci crede e ci tiene, è salva. La cordata di imprenditori italiani che la dovrebbe rilevare è ancora oscura e ancora non si sa chi sono coloro che la costituiranno. Carlo Toto, l'imprenditore abruzzese proprietario di Air One, non tirerebbe fuori un euro ma conferirebbe opzioni su un certo numero di *airbus* e poi la sua azienda, che non ha mai prodotto utili. I debiti al 31 dicembre 2007, inclusi i *leasing* degli aeromobili, superano i 200 milioni; il patrimonio netto, secondo la valutazione commissionata al perito di Chieti, è di 900 milioni. Se però si applicassero alla sua società i criteri di valutazione che si applicano alle compagnie aeronautiche il valore, tenendo conto dei debiti, non superebbe i 100 milioni. Come dire che un topolino comprerebbe un elefante. Vedremo. Certo è che Alitalìa è inserita in un contesto dove manca un piano generale dei trasporti. Vuol dire che ognuno fa un po' quel che gli pare. Sempre in quella puntata di «Report» è stato ricordato che a Siena vogliono ampliare il piccolo scalo di Ampugnano e farlo diventare un grande aeroporto per traffico internazionale. A pochi chilometri di distanza c'è un altro piccolo scalo civile, quello di Grosseto, e anche lì vorrebbero ingrandirsi, mentre a soli 100 chilometri di distanza ci sono gli aeroporti di Firenze e Pisa che da soli sarebbero sufficienti a coprire il traffico regionale. A Roma, oltre a Fiumicino, c'è Ciampino: la pista è a poche centinaia di metri dalle case e il traffico civile in aumento. Lo trasferiranno, forse a Viterbo. Nella pianura padana c'è un aeroporto ogni 50 chilometri, perché ognuno vuole il suo sotto casa, anche se è in perdita. Intorno a Malpensa ce ne sono addirittura una decina. Gli aeroporti sostituiscono gli investimenti nelle strade e nella rete ferroviaria o il servizio navetta che collega i maggiori aeroporti. Sono 45 gli scali aperti al traffico civile commerciale. Signor Presidente, civile commerciale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia dei Valori voterà a favore di questo decreto-legge per senso di responsabilità, ma sarà vigile per evitare che il buco nero di Alitalia continui ad allargarsi. Vogliamo un nuovo piano nazionale degli aeroporti, la liberalizzazione degli *slot*, ossia i diritti di decollo ed atterraggio, che limitati per legge non consentono ulteriori ingressi ad altre compagnie per avviare tiepide pratiche di concorrenza. Non siamo contro l'italianità, signor Presidente, onorevoli colleghi, e non abbiamo pregiudizi verso cordate italiane, purché vengano presentati piani industriali credibili, che consentano il risanamento di Alitalia e non il risanamento delle esposizioni bancarie degli acquirenti, di cui è costellata la storia di questo Paese. Vorremmo, inoltre, la salvaguardia dei posti di lavoro,

signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire brevemente in questo frangente esclusivamente per sottolineare quanto già espresso la scorsa settimana in occasione del voto di fiducia al Governo. In quella circostanza ho preannunciato che oggi avremmo approvato il cosiddetto prestito ponte nei confronti di Alitalia. Ribadisco che il prestito viene da noi approvato in quanto atto dovuto

la questione che ci sta veramente a cuore, per la quale, come Lega Nord, abbiamo lanciato il grido di allarme ancora nell'autunno scorso, largamente inascoltati, finché in campagna elettorale, come già ricordato da altri oratori prima di me, tutti sono diventati paladini del futuro dell'aeroporto di Malpensa. Ma ricordo perfettamente, avendo all'epoca ricoperto la carica di segretario provinciale della Lega Nord di Varese, la grande manifestazione tenutasi a Malpensa; solo di fronte ad essa l'opinione pubblica si è mobilitata e tutti hanno dovuto realmente prendere atto della situazione. Credo sia doveroso portare portare a conoscenza dell'Aula alcuni numeri inerenti ad Alitalia e Malpensa, al fine di fare chiarezza sulla differenza tra le due realtà. Storicamente i voli settimanali di Alitalia su Malpensa erano 1.236. Il taglio è stato di 886, con un residuo di soli 350 voli. Ma nel giro di un mese la semplice possibilità determinata da alcuni *slot* lasciati liberi ha permesso un recupero di 279 voli sugli 886, tagliati semplicemente in spregio alle necessità di mercato della zona. La situazione di questi tagli poc'anzi descritta ha determinato il prepensionamento di 310 unità, la collocazione in cassa integrazione di altri 900 operatori, senza tener conto degli esuberi dell'indotto, che ammontano a 2.500 unità accertate solamente per le aziende collegate all'attività di scalo di Malpensa, a cui si aggiungerebbero altri 6.000 esuberi, di cui circa 3.270 da aziende operanti nei comuni limitrofi all'aerostazione e circa 990 in altri settori (in prevalenza, ovviamente, il terziario). Tornando, invece, ai numeri di stretta competenza Alitalia, va rilevato che dopo l'abbandono di Malpensa le perdite da parte della compagnia di bandiera sono passate, dal consolidato milione di euro al giorno agli attuali 3 milioni di euro al giorno, esclusivamente a causa di quella forzatura del governo Prodi e dello sciagurato preaccordo con Air France. In questo, senatrice Bonino, i nostri pareri sono, ovviamente, diametralmente opposti. Peraltro, questo accordo con Air France

presa la decisione sul futuro di Alitalia (che molto poco interessa il territorio circostante Malpensa), si passi alle decisioni in merito al futuro destino del principale - non per principio preso, senatore Lannutti, ma per valenza statistica - aeroporto intercontinentale della Nazione. Approviamo, dunque, il prestito ponte per Alitalia; prendiamoci qualche mese per riflettere sul futuro della compagnia aerea, ma successivamente o sarà emersa una cordata di investitori seri in grado di inquadrare managerialmente la problematica e risanare l'azienda, oppure semplicemente dovremo dismettere Alitalia, chiudere una volta per sempre il buco nero di bilancio *(**Applausi dal Gruppo LNP)* a carico dei contribuenti padani e lasciare liberi gli spazi aerei di Malpensa per permettere ad altre compagnie serie e produttive di occupare un mercato innegabilmente presente sul nostro territorio.

in accoglimento della proposta avanzata in apertura di seduta dal senatore Zanda e condivisa da altri senatori, mercoledì 28 maggio, alle ore 9,30, la Presidenza svolgerà una Commemorazione solenne della figura di Aldo Moro, in occasione del 30° anniversario del suo assassinio e della strage della sua scorta per mano delle Brigate rosse. Potranno poi intervenire i rappresentanti dei Gruppi per quindici minuti ciascuno.

Per il momento, il Governo non dice: questo è grave, molto grave. È chiara la natura di questo provvedimento. Credo sia utile ripetere qui, di fronte al Parlamento,

Qui c'è un Governo che è in carica per gli affari correnti e c'è l'aspettativa di un Governo che, nella persona di colui che probabilmente lo presiederà, ha contribuito a far sì che la soluzione di Air France tramontasse, perché convinto di poterne proporre una migliore. È la bontà di questa proposta alternativa che giustifica l'atto di responsabilità di non far venir meno questa possibilità in questo momento». Vi è la responsabilità chiara dell'attuale maggioranza di aver reso impossibile l'accordo sulla soluzione Air France, sostenendo e legittimando le posizioni più conservatrici di una parte delle rappresentanze sindacali, rendendo chiaro all'offerente che, in caso di vittoria elettorale, il Governo entrante non avrebbe fatto fronte agli impegni derivanti da quell'accordo.

Ora, perciò, sta al Governo, che nella fase transitoria ha impedito il concretarsi di una soluzione e si è caricato di questa responsabilità, dimostrare di essere in grado di proporre una soluzione migliore una soluzione migliore sul piano delle alleanze strategiche, del servizio alla comunità nazionale e della capacità di creare ricchezza e perciò un'adeguata salvaguardia dei livelli occupazionali. Solo un'azienda sana e competitiva è in grado di dare certezze occupazionali. La retorica della compagnia di bandiera serve poco, molto poco. In un mercato del trasporto aereo globalizzato, la migliore difesa degli interessi nazionali si realizza con una società capace di competere alla pari nell'assicurare servizio e collegamenti. Compagnia di bravura, prima che compagnia di bandiera. Si è detto che il provvedimento è un decreto ponte, ma ponte verso che cosa? Questo non è un interrogativo banale, è un interrogativo sostanziale, a cui il Governo ha il dovere di dare una risposta, perché tempo non ce n'è più. I dati di gestione di Alitalia, li ha ricordati il senatore Legnini, registrano per il primo trimestre una perdita di 215 milioni di euro, con un crollo dei dei ricavi di oltre quattro punti percentuali. Con quali risorse potrebbe Alitalia far fronte agli oneri di questo prestito? E perché il prestito sia compatibile con i profili comunitari, occorre che la Commissione possa accertare con ragionevole certezza che l'operazione sarebbe accettabile da un investitore che opera in un'economia di mercato. È evidente che queste condizioni oggi non ci sono, perché quel ponte, appunto, dall'attuale Governo non è stato costruito. si è accusato il passato Governo di essere giunto alla scelta della proposta di Air France con un percorso non trasparente. Nulla di più falso! Ricordo che, tra dicembre 2006 e luglio 2007, si svolse una apertissima procedura competitiva, con 11 manifestazioni di interesse, tre successive offerte preliminari, ma nessuno dei concorrenti giunse a presentare un'offerta vincolante. Nella seconda fase, fu invitata Alitalia all'individuazione di soggetti industriali e finanziari interessati all'operazione. Di 28 soggetti interessati, sei furono ammessi alla prosecuzione alla prosecuzione delle trattative e due presentarono offerte vincolanti. Infine Alitalia, d'intesa con il Governo, decise la trattativa in esclusiva con Air France. Questa fu la procedura, allora. Ed oggi? L'unica cosa che l'opinione pubblica e il Parlamento sono in grado di sapere è che il finanziere Bruno Ermolli, definito sulla stampa consulente di Silvio Berlusconi, sta lavorando alla definizione di una cordata. Non si sa attraverso quali procedure, quali organi di valutazione e quali momenti di confronto competitivo il Governo intenda concludere l'operazione Alitalia. Noi voteremo a favore di questo decreto. Lo facciamo per atto di responsabilità verso l'azienda, i suoi dipendenti e verso gli interessi nazionali, ma non possiamo non registrare che il Governo viene meno alle sue responsabilità, quella di presentare oggi, se non la soluzione almeno un percorso chiaro per arrivare alla soluzione nei tempi ristrettissimi che la situazione così difficile consente.

*(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia dei Valori esprime il proprio assenso alla conversione in legge del decreto sull'erogazione di un prestito in favore di Alitalia. Dopo le perplessità manifestate in precedenza, questa volontà è maturata e si è consolidata in considerazione soprattutto della preoccupante situazione in cui si è venuta a trovare la nostra compagnia di bandiera. Una situazione che tutti noi ormai conosciamo e che presenta anche aspetti drammatici, come dimostrano le giuste aspettative dei lavoratori della compagnia e dell'indotto, messe a dura prova dall'incertezza sul futuro dell'azienda. Rendendosi conto di ciò, il precedente Governo non ha mancato di cercare, seppur affannosamente, soluzioni o interventi che potessero procrastinare il precipitare degli eventi. In tale condizione, il Governo Prodi, emanando questo decreto che ha portato all'erogazione del prestito di 300 milioni di euro, ha inteso dare respiro alla società e speranza ai lavoratori, dilazionando in qualche modo le urgenze, per consentire poi al nuovo Governo le più opportune valutazioni. un prestito che ricordiamo essere stato concesso secondo modalità ben definite per quanto riguarda la restituzione del capitale, come evidenziato dall'articolo 1, Noi dell'Italia dei Valori ribadiamo che il nostro parere favorevole alla conversione in legge del decreto in esame è una dimostrazione di responsabilità, un atto consapevole di continuità con quanto fatto e sostenuto anche dal presidente Antonio Di Pietro nel Consiglio dei ministri del precedente Governo. Dunque, è soltanto per un forte senso di responsabilità che mostriamo la nostra disponibilità, non certo perché sollecitati da chi nell'ultima campagna elettorale ha utilizzato la grave crisi di Alitalia a fini puramente speculativi e propagandistici. Ora che abbiamo potuto constatare come la cordata annunciata dall'attuale Presidente del Consiglio sia in realtà una chimera, non possiamo che ribadire la nostra speranza. Oggi, in un momento oltremodo delicato, che non va sottovalutato e che richiede coscienza intellettuale e morale, auspichiamo che questi soldi vengano ben utilizzati, per mantenere costante il livello di attività di Alitalia e il pieno funzionamento del servizio, con l'accortezza di non incidere sulla vita di migliaia di lavoratori e relative famiglie, evitando provvedimenti restrittivi e tagli ingiustificati. Nell'attesa, certamente non più procrastinabile, che si possa finalmente risolvere la questione attraverso una formula soddisfacente, soltanto ventilata dal nuovo Governo, ci auguriamo una soluzione che guardi all'italianità, alla tradizione ed alla storia della compagnia e che sappia coniugare l'efficienza del trasporto aereo con i giusti profitti, ma soprattutto con il mantenimento, il rafforzamento e la sempre più alta qualificazione dell'attuale forza lavoro. Noi dell'Italia dei Valori riteniamo, inoltre, che queste considerazioni non debbano essere disgiunte dalla necessità di tenere sempre presente l'importanza della sede di Malpensa, nodo strategico della Lombardia e dell'intero Nord Italia, che ha valide motivazioni di esistere e che può ritrovare impulso e sviluppo soprattutto di fronte alla sfida internazionale che ci attende da qui a sette anni e che ci riguarda tutti, l'Expo di Milano del 2015, nel quale confidiamo per il rilancio della nostra economia. *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione odierna sul decreto relativo al prestito ponte di 300 milioni di euro si colloca in un contesto di acuta drammaticità per la nostra compagnia di bandiera. Nonostante l'allarme sui conti duri da tempo, l'impegno a ridurre i costi non è approdato a nulla, anzi, la situazione peggiora a vista d'occhio e l'emergenza si aggrava. Il primo trimestre 2008, confrontato con il primo trimestre 2007, vede salire la perdita prima delle imposte a 215 milioni, ben 62 milioni in più rispetto all'esercizio precedente. di Alitalia indica i principali motivi del peggioramento nel caro petrolio, contro il quale però - voglio rimarcare - Alitalia non ha copertura assicurativa, contrariamente alle altre principali compagnie aeree, di amministrazione - «nell'erosione della credibilità commerciale (...) con rilevanti ripercussioni sullo sviluppo delle vendite e la riduzione di traffico determinate dalla modifica del *network*». Fuori dalle parole paludate del consiglio di amministrazione, c'è stato un calo pesante di passeggeri. Gli italiani volano sempre di più, ma sempre di meno con Alitalia. Il traffico è infatti raddoppiato negli ultimi 7-8 anni con il contributo anche delle *low cost*. Nel 2007 i passeggeri sono stati 82 milioni; Alitalia rimane inchiodata a 25 milioni di passeggeri. Al 31 marzo 2008 il patrimonio netto ammontava a 360 milioni, in caduta libera dai 573 milioni di fine 2007. Ecco perché senza il prestito ponte di 300 milioni, oggi - com'è stato rimarcato da altri colleghi - la compagnia sarebbe vicinissima al fallimento. Di più: al ritmo di quasi tre milioni al giorno di perdita, tutti siamo in grado di calcolare in massimo 100 giorni l'ossigeno che resta e il *countdown* è già cominciato. Ma senza una prospettiva rischiamo solo di bruciare altri soldi dei contribuenti italiani. Se questo è il quadro, drammatico, credo che si debba essere molto chiari e molto netti nel chiedere al Governo Berlusconi certezze sul futuro di Alitalia. Noi responsabilmente voteremo il decreto-legge in esame, ma proprio per questa ragione siamo ancora più netti nel chiedere risposte al Governo. Com'è noto, il Governo Prodi, di fronte alla china pericolosa della compagnia di bandiera, aveva avviato responsabilmente un percorso di privatizzazione, culminato nella proposta di Air France, proposta da tutti gli analisti giudicata seria, capace di risolvere non solo i contingenti guai finanziari, ma di dare una prospettiva futura ad Alitalia, con un piano industriale che comportava certo anche sacrifici, ma in grado di legare stabilmente Alitalia al più grande *network* di trasporto aereo del pianeta e quindi in grado di definire un quadro di certezze per gli utenti e per i lavoratori. Questa proposta è stata ritirata a seguito delle polemiche elettorali del centrodestra, all'insegna della difesa di una malintesa italianità della compagnia. Si è detto no ad Air France, anche in nome del Nord, della difesa di Malpensa. Ad oggi il risultato è che alla crisi di Alitalia si è aggiunto l'abbandono di Malpensa al suo destino (noto che anche gli amici della Lega sono molto più morbidi nella difesa del Nord e di Malpensa). dopo i proclami e le manifestazioni della Lega sono giunte proposte serie sul futuro dello scalo milanese, che appunto sta facendo da sé. Dalle parole dei colleghi della Lega questo emerge; nessuna proposta da parte del Governo Berlusconi. Il presidente Berlusconi ha evocato in questi mesi più volte una cordata italiana in grado di acquistare Alitalia, cordata che è l'oggetto misterioso che riempie le pagine dei giornali. Ma a me, che piace anche la vita di Internet, sembra più una creatura di *Second life*, una mera realtà virtuale, non una seria proposta finanziaria e industriale. di Alitalia non ha potuto far vedere i conti al superconsulente ragionier Ermolli per la semplice ragione che la fantomatica cordata Ermolli non ha presentato ad oggi alcuna offerta di privatizzazione di Alitalia e quindi la *due diligence* non è ovviamente possibile, perché il signor Ermolli è ad oggi un privato cittadino e nulla più. Il dibattito odierno deve quindi fare chiarezza in modo definitivo. Ricordo - è già stato indicato dalla collega Bonino - che la *condicio* *sine qua non* per considerare il prestito ponte fuori dal campo di applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato era in primo luogo che vi fosse un acquirente certo, in secondo luogo che l'erogazione fosse conclusiva per l'operazione. Queste condizioni erano soddisfatte dalla proposta di Air France. Qualunque proposta alternativa deve fare altrettanto, pena la censura europea. Perqueste ragioni chiediamo che il Governo indichi di fronte al Parlamento quale soluzione dare alla crisi di Alitalia, oggi o possibilmente - se non oggi - nelle giornate successive, ma non si può dilazionare a lungo una risposta al Parlamento da parte del Governo. Questa risposta la dobbiamo agli utenti, che ancora seguono Alitalia, sia pure in numero sempre minore; la dobbiamo ai lavoratori, che vedono il proprio posto di lavoro minacciato (ricordiamo le manifestazioni dei dipendenti qualche settimana fa); la dobbiamo ai contribuenti italiani, che in dieci anni hanno dato ad Alitalia una cifra astronomica, qualcosa come 5 miliardi di euro. Il Governo quindi deve indicare qual è il partner finanziario, qual è il partner industriale che pensa per Alitalia. Il tempo è ormai ampiamente scaduto. Se non verranno risposte chiare, se non verranno risposte rapide, non resterà altro che la strada del commissariamento. I cittadini e i lavoratori sapranno di chi è la responsabilità.

ha fatto investimenti ed ha mantenuto la compagnia di bandiera per tanto tempo, mentre da Roma si è sempre risposto contro questo modo di operare.

di non metterla in vendita*tout court* ma di cercare eventualmente il compratore. Penso sia quello che il Presidente del Consiglio ha annunciato durante la campagna elettorale e che mi auguro vada a buon fine. Il compratore, però, non deve essere

di industriali. Suggerirei di prevedere una quota di azionariato popolare in modo che gli abitanti, i residenti, i cittadini italiani

Vorrei anche che si lasciassero liberi gli *slot*. Non vorrei che la compagnia di bandiera, in una situazione di ristrutturazione, non liberasse gli *slot* di Malpensa, mettendo fortemente in difficoltà

Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare il relatore, che ha dato conto del dibattito in Commissione in maniera precisa e puntuale. Voglio subito aggiungere, rivolgendomi al rappresentante del Governo, che mi ha impressionato la posizione del Governo espressa in Commissione. Sostanzialmente si chiede tempo per trovare una soluzione ad un problema che si dichiarava essere risolto o risolvibile nel giro di poco tempo a patto che il Governo uscente desse la possibilità a quello entrante di guadagnare qualche giorno di tempo attraverso un decreto‑legge apposito ed un prestito ponte per dar corpo ad una iniziativa che avrebbe messo in campo una cordata già presente, già operativa, già in grado di rilanciare il futuro industriale dell'Alitalia. Purtroppo oggi prendiamo atto, anche dalle dichiarazioni rese in quest'Aula e dagli interventi dei rappresentanti della maggioranza, che quella soluzione non c'è e che è da ricercare,

in relazione agli impegni precedentemente assunti e tesi alla privatizzazione dell'azienda di trasporto aereo in un quadro di rispetto delle norme comunitarie. Vorrei aggiungere che il problema Alitalia non nasce oggi, visto che sembrerebbe che l'Aula approcci questo problema per la prima volta. Il Parlamento e il Governo si sono occupati di Alitalia in più circostanze. Per esempio, nel 2002, quando fu disposto un incremento di capitale di circa 900 milioni di euro con un provvedimento motivato dall'obiettivo di promuovere un piano di ristrutturazione e di rilancio dell'azienda. Il Parlamento e il Governo si occuparono di Alitalia due anni dopo, nel 2004, quando fu discusso e approvato il decreto-legge n. 159, che offriva garanzie dello Stato su un prestito ponte (anche quello fu definito prestito ponte) di 400 milioni di euro

che furono risolte attraverso una procedura rituale e formale che si sostanziò in un atto di impegno, sottoscritto dal Ministro per le politiche comunitarie in data 13 13 luglio 2004, che si impegnava ad agire senza disporre ulteriori interventi da parte dello Stato (ulteriori aiuti di Stato) entro i 12 mesi dalla concessione del prestito ponte, cioè dal luglio 2004. del Senato discusse la conversione di quel decreto il 14 luglio e il titolo, ancora una volta, era relativo a misure urgenti per favorire la ristrutturazione e il rilancio di Alitalia. Per curiosità ho voluto leggere i resoconti di quel dibattito parlamentare e ho avuto l'impressione che i senatori allora parlassero per oggi, o che oggi parlino per allora, perché i termini del problema non sono affatto modificati, le questioni rimangono tutte tutte valide, le valutazioni espresse allora sono state riconfermate in questa sede, il Governo annuncia gli stessi impegni che furono annunciati nel 2004. è una sola differenza rispetto ad allora: cambiano i numeri che sostanziano quei giudizi, cambiano i numeri in riferimento alle perdite,

circa la riduzione del fatturato, del traffico effettivo, della capacità complessiva, del fattore di riempimento. I numeri di oggi dicono che Alitalia rischia una situazione di non ritorno; ci dicono che il tempo a disposizione è scaduto, e il tempo non lavora per Alitalia. Giova infatti ricordare che, mentre Alitalia si impoverisce, mentre Alitalia abbandona quote di mercato, mentre Alitalia perde *appeal* rispetto ai consumatori, ai quali non riesce a conferire quel valore aggiunto dato dalla sicurezza offerta da un grande operatore nazionale, altri operatori si rafforzano, altri operatori recuperano, occupano lo spazio lasciato libero Questa situazione vorrei che venisse relazionata alla presunta tutela dell'interesse nazionale, che evidentemente passa in secondo piano. una spirale che va bloccata, che va interrotta, perché le soluzioni che oggi appaiono onerose domani appariranno come le soluzioni auspicabili, quelle per le quali sarà necessario concentrare il massimo degli sforzi affinché si possano realizzare. Il dibattito del 14 luglio 2004 è emblematico. Immagino che il collega Cicolani avrebbe oggi replicato l'intervento fatto esattamente quattro anni fa in quest'Aula. Disse allora: «Vi sono stati errori commessi nel passato e non mi interessa dire se dal centrodestra o dal centrosinistra». Mi preme sottolineare che sono stati commessi degli errori. E aggiungeva: «Il processo di privatizzazione e il tentativo fallito di accordo con la KLM tre anni fa oggi avrebbero consentito di avere una compagnia di dimensioni maggiori, quindi con una massa critica maggiore e con una forza finanziaria maggiore, che avrebbero consentito di muoversi da quel punto morto in cui si trova l'Alitalia, che è talmente grande da essere condizionante nel sistema economico del nostro Paese» - ecco l'interesse nazionale - «ma purtroppo ancora troppo piccola per poter conseguire quella politica di rilancio che permetterebbe in parte di affrontare dalla parte dei ricavi

e aveva assunto impegni vincolanti con la Commissione europea; e solo in ragione di quegli impegni fu varato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2005, recante modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia in Alitalia, che rappresentò l'atto conclusivo di una vicenda piuttosto controversa. Ed è in ragione di quelle procedure che si era giunti qualche mese fa alla soluzione. Esisteva una soluzione che avrebbe tutelato gli interessi nazionali, che avrebbe salvaguardato la compagnia di bandiera, che avrebbe messo il nostro Paese nella condizione non solo di conservare, ma di accrescere il proprio posizionamento competitivo nel trasporto aereo. Certo, ciascuno di noi avrebbe voluto che quelle soluzioni fossero... *(Il microfono si Ma quelle soluzioni erano obbligate in ragione della situazione che si era determinata.

nei tempi richiesti dal mercato, nei tempi richiesti dalle logiche industriali che presidiano questi settori.

ponte di breve termine alle condizioni di mercato e della durata strettamente necessaria, tanto che dovrà essere restituito entro il 31 dicembre 2008 ed è gravato anche di un tasso d'interesse di mercato.

400 milioni di euro con la garanzia dello Stato. Credo che avremmo dovuto perseguire quello stesso obiettivo, anche alla luce di quanto è emerso dalle osservazioni del Servizio bilancio. Cerchiamo di superare

per due anni siete stati al Governo; certo, ci siamo stati anche noi dal 2001 al 2006, ma la situazione si è aggravata nell'ultimo periodo. Meno male, Meno male, collega Bubbico, che siamo intervenuti a bloccare la svendita - che volevano Prodi e il ministro Padoa-Schioppa e probabilmente non la maggioranza che non aveva approfondito questo aspetto - all'Air France-KLM. Anche

allora con un distinguo e motivazioni diverse. Dobbiamo individuare un partner che sia capace di dare veramente una soluzione al problema dell'Alitalia. Noi stessi, probabilmente, come cittadini, dobbiamo renderci conto della necessità dell'esistenza dell'Alitalia, che è una bandierina piantata in tutto il mondo e che sviluppa

quando entreremo nello specifico, quando il Governo avrà individuato una proposta concreta e la offrirà all'esame e al dibattito: in quella sede potremo essere più precisi.

così come ci veniva suggerito anche dalla Commissione europea. Accingendomi a concludere questo mio intervento e preannunciando il voto favorevole del Gruppo del del Popolo della Libertà, ferme rimanendo le preoccupazioni che abbiamo sull'avvenire dell'Alitalia, confidiamo però nell'azione del Governo del presidente Berlusconi affinché possa trovare una soluzione idonea che sappia coniugare

Esprimo ancor più convintamente l'apprezzamento per il fatto che, nonostante alcune corrette osservazioni critiche, da parte dei Gruppi si è ribadita l'intenzione di votare a favore della conversione di questo decreto-legge che a noi pare assolutamente essenziale. Nella mia brevissima replica desidero recuperare poche osservazioni per aggiungere schematicamente alcune cose a quanto già detto in Commissione. Al collega Legnini voglio ricordare che, è vero, il Ministro in Commissione non è venuto, ma, come abbiamo avuto modo di spiegare, proprio ieri era impegnato in un incontro con le rappresentanze sociali per illustrare in un confronto aperto i provvedimenti che sarebbero

un finanziamento ponte. Non vorrei che sul nominalismo di alcune affermazioni ci dividessimo, quasi a spezzare il capello in due. Questo è un finanziamento che a data certa deve essere restituito, che non incide sui saldi di finanza pubblica e che, quindi, non modifica gli equilibri di bilancio. Libertà nostra di considerarlo a tutti gli effetti un finanziamento ponte, libertà vostra di dire che non lo è e che è qualcosa di diverso che non si sa come definire. Nella sostanza, questo è un finanziamento

scoprire le carte e dire come intende procedere. Alla collega Bonino, con tutta la benevolenza, il rispetto e la stima

lasciamo che i giornali si sbizzarriscano immaginando che in Parlamento ci siano un partito che tende a difendere l'italianità e un altro che non l'ha a cuore. Credo che questo non sia un problema. peraltro, non ho l'ambizione di essere l'interprete autentico del pensiero del Governo Berlusconi. molto difficile per il relatore svolgere il suo intervento e per chi vuole, ascoltarlo. Vi prego di tenere comportamenti che consentano un dibattito in situazioni normali e istituzionalmente corrette. Si può chiacchierare fuori,

Sgombrato il campo da questo equivoco tutto di stampo massmediale, vediamo di curarci più del merito delle questioni. Ritengo che il Governo Berlusconi si sia mosso nella convinzione di due punti di riferimento precisi.

Italia. La settima potenza mondiale sul piano economico ha inoltre bisogno di tutelare i suoi interessi nel settore logistico e trasportistico e io non credo che possa farlo al meglio immaginando di essere mediata da una compagnia incorporata da un'altra compagnia straniera. In ultimo, signor Presidente, mi creda, qui le bandiere non c'entrano,

che Governo e Parlamento, nel rispetto delle leggi esistenti e delle direttive comunitarie, sappiano curare e difendere gli interessi del nostro Paese.

i presidenti Prodi e Berlusconi hanno giudicato dovesse essere approvato per evitare, questo sì, il tracollo di una situazione che, probabilmente,

privatizzazione di Alitalia è quello di fornire al sistema Italia un sistema competitivo in grado di servire al meglio gli italiani e le loro merci, ai prezzi più convenienti possibili. Questo è, in sostanza, l'oggetto di questo decreto-legge. Ricordo che si tratta di un oggetto molto limitato non si tratta dell'esaurimento della pratica della privatizzazione di Alitalia o della soluzione del problema del trasporto aereo, ma semplicemente di costituire una sorta di ponte tra il vecchio e il nuovo.

visto quanto recita il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge: «La somma erogata ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione dell'intera quota del capitale sociale,

l'ultimo e unico meccanismo che consente di attuare la politica che tutti desideriamo in materia di trasporto aereo. Un'ulteriore precisazione concerne la preoccupazione che il prestito si configuri come aiuto di Stato. In realtà si tratta di una mera anticipazione finanziaria reversibile, con caratteristiche di mercato a brevissimo termine a valere sui fondi di tesoreria. Per inciso, i fondi di tesoreria che vengono attivati sono quelli del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, che ha una capienza assolutamente sufficiente e che comunque verrà

assicurare che il Governo è disponibile a presentarsi nella sede che il Senato riterrà più opportuna per discutere il futuro dell'Alitalia e chiedere all'Assemblea la sollecita conversione di questo importante decreto-legge.

siamo chiamati ad esaminare un decreto-legge che prevede un finanziamento ponte da 300 milioni di euro ad Alitalia al fine di garantire, per un periodo di tempo limitato ossia strettamente necessario, un servizio pubblico essenziale ed evitare problemi di ordine pubblico. Tutti sappiamo che il finanziamento ponte nasce da un'intesa *bipartisan*; è stato erogato lo scorso 5 maggio in base al decreto-legge del 23 aprile del Governo Prodi concordato con Silvio Berlusconi, al fine di garantire alla compagnia di bandiera la sopravvivenza. Entrambe le Camere dovranno approvare il succitato decreto entro il prossimo 23 giugno, pena la decadenza. La Commissione speciale addetta alla conversione dei decreti-legge, di cui sono membro, ha trasmesso il testo a quest'Assemblea dopo un attento esame dello stesso. Tale intervento, come si legge nella relazione del provvedimento, si reputa necessario ed urgente in considerazione della gravissima situazione finanziaria di Alitalia, ben nota a noi tutti. Sappiamo che la situazione finanziaria della compagnia aerea si è aggravata anche a causa del caro petrolio.

grazie a questo finanziamento ponte, che fortunatamente non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica né variazioni di bilancio. Infatti, il decreto-legge prevede che il prestito dovrà essere rimborsato entro la fine di quest'anno. In Commissione, in corso di esame, sono stati espressi vari dubbi sul provvedimento, soprattutto sui suoi profili comunitari: uno dei rischi che corriamo è quello di una sua bocciatura da parte della Commissione europea, qualora l'Unione Europea considererà questo finanziamento come un aiuto di Stato, visto che il decreto-legge è firmato dal Ministro dell'economia azionista di Alitalia. Ora non intendo entrare nel merito della legittimità del provvedimento, fatto sta che le perdite di Alitalia vengono stimate a quasi tre milioni di euro al giorno e che, allo stato, la tanto evocata cordata italiana non esce allo scoperto. Onorevole Presidente, cari colleghi, vista la rinuncia di Air France il tempo di strutturare ed organizzare eventuali soluzioni alternative si fa sempre più stretto. Occorre risolvere tale questione positivamente e definitivamente, tenendo conto dell'interesse nazionale, ma nel rispetto delle regole del mercato. Per rendere questo Paese più moderno ed efficiente e per rilanciare la nostra economia servono infrastrutture ed un buon sistema di trasporti. Ma occorre trovare in tempi brevi una soluzione alla crisi di Alitalia, soprattutto perché non è più tollerabile che a pagare i conti in rosso di questa compagnia siano i nostri cittadini, che hanno urgentemente bisogno di risposte concrete in campo economico e sociale. Onorevole Presidente, annuncio che i membri del Gruppo UDC, SVP e Autonomie esprimeranno liberamente il loro voto secondo le proprie convinzioni. Posso tuttavia preannunciare che i miei colleghi Helga Thaler Ausserhofer, Oskar Peterlini, Mirella Giai, Antonio Fosson ed io esprimeremo voto favorevole al provvedimento in esame.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, con il provvedimento al nostro esame viene disposto in favore di Alitalia S.p.A. il cosiddetto prestito ponte di 300 milioni di euro, a valere su fondi di Tesoreria, senza tuttavia - come spiega la relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge - comportare effetti sui saldi di finanza pubblica, né variazioni di bilancio. Infatti, i fondi erogati dalla Tesoreria verranno ricostituiti alla restituzione del prestito, maggiorati degli interessi maturati. Si stabilisce, inoltre, che il prestito verrà rimborsato entro il 31 dicembre 2008, maggiorato di un tasso di interesse nella misura prevista dalla specifica disciplina comunitaria richiamata. Si dispone quindi che, fino al rimborso del prestito ponte, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'Italia sono equiparati a quelli *ex* articolo 67, comma 3, lettera *d)*, della legge fallimentare. Appare evidente che il prestito in favore di Alitalia S.p.A. si rende necessario ed urgente in seguito alla gravissima situazione finanziaria della stessa società, per far fronte all'immediato fabbisogno di liquidità dell'azienda, anche al fine di garantire una continuità dell'attività ordinaria nel breve periodo. Per questo motivo, signor Presidente, voteremo a favore del presente disegno di legge. Tuttavia, dobbiamo esprimere alcune perplessità in merito alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato alle imprese del prestito concesso dal Governo ad Alitalia. L'assenza di un piano industriale rafforza l'ipotesi di un prestito al limite della compatibilità con le norme comunitarie. Secondo la giurisprudenza comunitaria, infatti, gli incentivi alle imprese in difficoltà, per essere dichiarati compatibili con il mercato comune, devono accompagnare un piano di ristrutturazione coerente, che deve essere presentato alla Commissione europea con le necessarie precisazioni. Nel caso del prestito ponte ad Alitalia, invece, nonostante l'opposizione abbia sollecitato sia il Governo, nella persona del Ministro dell'economia, sia i vertici aziendali ad intervenire per spiegare meglio quali siano i loro orientamenti sul futuro dell'azienda, allo stato attuale dobbiamo registrare con grande rammarico che non esistono né un piano industriale, né le necessarie motivazioni, a parte l'affermazione secondo cui il contributo, considerate le ragioni di ordine pubblico e l'urgenza della situazione finanziaria, dovrebbe garantire la continuità del servizio a favore degli utenti. In particolare, i motivi di ordine pubblico non sembrano decisivi. Infatti, non solo la normativa comunitaria non prevede, almeno in generale, l'ammissibilità di aiuti di Stato

se non vi ha contribuito, ha specifiche responsabilità. Vale la pena di ricordare che nel 2002 il bilancio di Alitalia è risultato positivo per 93 milioni di euro; nel 2003 si è avuta una perdita di 520 milioni di euro, saliti a 844 l'anno successivo; nel 2005 la perdita è stata contenuta a 168 milioni, per poi risalire nel 2006 a 605 milioni di euro e fermarsi nell'ultimo bilancio annuale del 2007 a 364 milioni di euro. Fino ad oggi, quasi tutte le perdite sono state a carico dello Stato. Si parla di un buco di gravità enorme, considerando anche i periodi non citati. Alla fine del 2006, il Governo Prodi è stato costretto all'ennesima ricapitalizzazione, decidendo di vendere la compagnia al miglior offerente. Si sono formate una decina di cordate, ma tutte alla fine hanno rinunciato, giudicando troppo vincolanti e impraticabili le condizioni imposte per il compratore. Nell'estate del 2007 si è deciso di andare a trattativa privata e, per limitare le spese, si è elaborato un piano che prevede, tra l'altro, il taglio di 150 voli da Malpensa.

Ricordando ancora che nel 2003 si è avuta una perdita di 520 milioni di euro, saliti a 844 l'anno successivo, che nel 2005 la perdita è stata contenuta a 168 milioni, per poi risalire a 605 milioni nel 2006, e che il Governo Prodi è entrato in carica nella metà del 2006, l'Italia dei perché Silvio Berlusconi non abbia risanato la compagnia di bandiera quando era al Governo. Adesso egli afferma che o si fa l'Alitalia o si muore, facendo appello ad un improprio sentimento di italianità che costerebbe che costerebbe ai contribuenti un prezzo troppo alto. Ma i contribuenti ed i lavoratori di Alitalia hanno le tasche piene di promesse: oggi chiedono certezze, quelle certezze che l'attuale Governo, in questo momento, non ha saputo dare. Alitalia perde 3 milioni di euro al giorno, quindi il cosiddetto prestito ponte finirà in fretta. A quel punto, cosa succederà? Avremmo voluto sentire il Governo sul futuro dell'azienda di bandiera del nostro Paese. Il presidente del Consiglio Berlusconi, in campagna elettorale, ci aveva promesso la cordata, ma nessuno l'ha vista. Possiamo supporre che chiederanno ancora alle banche di intervenire per salvare Alitalia e per fare qualche cordata che altrimenti nessun imprenditore si sognerebbe di fare, perché evidentemente vorrebbe ricevere dei quattrini per comprarla e non certo metterci capitali freschi. Noi dell'Italia dei Valori esprimiamo quindi una viva preoccupazione perché in un Paese serio le trattative vanno condotte su altri presupposti, che rispondano alle esigenze del mercato, senza ricorrere ad una definitiva stabilizzazione della compagnia di bandiera. Il senso di responsabilità e la coerenza impiegati nel decreto‑legge approvato dal Governo di cui l'Italia dei Valori era partecipe non faranno mancare un voto favorevole, con l'esortazione al Governo di tenere un comportamento trasparente, non sottraendosi mai alle informative puntuali che il Parlamento gli chiederà. *(Applausi

prende la parola un esponente della Lega, indubbiamente tutti quanti, anche senza usare toni eufemistici, sanno che a parlare non è sicuramente una persona di carattere ultranazionalista. Oggi, però, ci dobbiamo confrontare proprio su un problema di carattere nazionale, ossia se salvare o meno la compagnia di bandiera. Si sa anche che, come Lega, amiamo molto più le bandiere regionali

Prendiamo atto di quella che è stata la storia di Alitalia e del fallimento dell'ultimo tentativo di vendita della quota di controllo

Abbiamo verificato cosa accade in caso contrario e abbiamo tirato delle conclusioni: non vi sono alternative a questo provvedimento; un eventuale parere negativo significherebbe il fallimento immediato della compagnia di bandiera. Qual è la speranza che anima probabilmente tutti quanti, noi compresi? È che da ora alla fine del 2008 si riesca a trovare un partner solido che sappia acquisire le quote di maggioranza che verrebbero cedute.

si sa che fanno incontri, tavoli di verifica; ci sono gruppi come Ligresti, Tronchetti Provera, Polegato, Fossati ed altri interessati a questa operazione.

sono le tipologie di aerei in dotazione di Alitalia. Nessuna compagnia ha fatto questa diversificazione; per lo più si opta per tecnologie *boeing* o tecnologie *airbus*. Alitalia ha diversificato acquistando - forse l'unica compagnia al mondo - anche aerei prodotti in Brasile: sotto la presidenza di D'Alema, infatti, si acquistarono degli *embraer* forse per fare un piacere al presidente Lula appena insediato. Si parlava di *partnership* industriali-economiche, ma di fatto si realizzavano delle *partnership* politiche con quei Paesi sulla pelle di Alitalia e di in Alitalia operava.Questo comunque è il passato. Oggi - abbiamo ascoltato l'intervento della collega Bonino - c'è chi obietta che la Commissione europea potrebbe anche bocciare questo provvedimento. Infatti gli orientamenti della Comunità, per lo più mercantilistici, perseguono effettivamente i fini di cui ha parlato la senatrice. L'uscita delle imprese inefficienti rientra nel normale funzionamento questi sono gli orientamenti della Comunità. Però la Comunità ha sempre smentito queste voci eccessivamente allarmistiche: ricordiamo che in occasione dell'ultima ricapitalizzazione di Alitalia, quando si divise la società

A questo punto ai colleghi che hanno qualche rimostranza dico che se quell'operazione al limite, molto *borderline*, fu giudicata nel contesto rispettosa e legittima, a maggior ragione un prestito, per lo più a termine, per lo più a tassi di mercato, non potrebbe oggi essere essere obiettato e sollevato. In ogni caso noi dobbiamo essere anche obiettivi, nel senso che non possiamo continuamente guardare a questa Europa come un'Europa matrigna; non possiamo concepire un'Europa che non ci consenta neanche in questo caso Non possiamo accettare un'Europa che ci dica che non possiamo produrre latte e poi ci obbliga a comperarlo all'estero a prezzi sempre più esagerati; come non possiamo accettare un'Europa che decide di far chiudere le nostre aziende perché non le sa difendere da una concorrenza sleale dovuta ad un'economia globale sregolata, per lo più indocinese. Sappiamo però che questo è un altro argomento. Sulla questione Alitalia, la Lega Nord è favorevole al prestito ponte, pertanto alla conversione del decreto-legge *(PD)*. Signor Presidente, il Partito Democratico voterà a favore della conversione del decreto-legge che autorizza il prestito all'Alitalia e lo farà nonostante un radicale dissenso dalle modalità irrituali, opache e anche rischiose con le quali l'onorevole Berlusconi nei mesi passati, ben prima essere capo del Governo, ha interferito sulla crisi dell'Alitalia e ora, con più titolo, la sta gestendo. Il Partito Democratico voterà il provvedimento per due motivi consistenti: per solidarietà nei confronti dei lavoratori di Alitalia e per dare atto al presidente Prodi della sensibilità istituzionale e politica di cui ha dato prova anche dopo il 13 aprile, emanando un decreto-legge che in ogni sua parte, dal dispositivo allo stanziamento, rispondeva alle indicazioni di Berlusconi.

e cioè che Silvio Berlusconi predichi bene, ma poi sia tentato di razzolare male: parla di garbo e di gentilezza, ma poi lui, fatto salvo qualche salamelecco superficiale, di garbo non ha alcuna intenzione di concederne nemmeno un'oncia. Insomma, ci sono molti segnali che Berlusconi con questa storia della gentilezza voglia cloroformizzare, confondere, in una parola intortare l'opposizione e se questa è la sua intenzione sappia che non ci riuscirà. Con la maggioranza colloquieremo sulle regole; sulle riforme avremo un atteggiamento politico costruttivo, molto diverso da quello che ha avuto il centrodestra nei 20 mesi di governo Prodi: è nostro dovere farlo e serve all'Italia. Ma non faremo sconti, né sul piano politico parlamentare, né sulle azioni di Governo. Se il presidente Berlusconi oggi fosse qui, gli avrei detto che meglio avrebbe fatto a parlare di lealtà e franchezza più che di garbo e gentilezza, perché, signori senatori - e mi rivolgo soprattutto ai senatori della maggioranza questo è il punto politico che caratterizzerà questa legislatura: i rapporti tra maggioranza e opposizione potranno evolvere in una direzione o in un'altra soltanto in relazione alla qualità del confronto e alla lealtà del dibattito di cui saremo capaci. Per risolvere i problemi gravi dell'Italia servono verità e lealtà, più che galateo televisivo. Purtroppo, quanto a qualità di contenuti la maggioranza non è partita con il piede giusto. Finora, sul caso Alitalia non abbiamo ascoltato alcuna franca analisi delle ragioni della crisi e alcuna chiara descrizione delle strategie e dei progetti per il futuro. La crisi dell'Alitalia - lo sapete - viene dalle degenerazioni degli anni Ottanta e Novanta, che hanno caratterizzato la nostra industria di Stato, anni di ampie e diffuse responsabilità della politica, del sindacato, del *management* e di tanti altri comprimari, ma la data che segna il passaggio da una condizione di difficoltà a un dramma aziendale è quella dell'11 settembre 2001. È dopo quella data che nessuno è rimasto come prima nel trasporto aereo mondiale, basti pensare all'immediata contrazione della domanda, all'aumento del costo del carburante, al rallentamento delle economie occidentali, alla necessità di aumentare la sicurezza negli aeroporti e all'emergere delle compagnie a basso costo. In tutto il mondo, dopo l'11 settembre, tutti hanno aperto gli occhi: i governi e le compagnie aeree; chi ha capito ha preso le contromisure, chi non ha capito ne sta subendo ancora le conseguenze. Sono quelli gli anni in cui Sabena e Swissair fallivano e si ristrutturavano, British entrava nell'azionariato di Iberia e tutte - dico tutte - le maggiori compagnie degli Stati Uniti cambiavano radicalmente pelle. In Italia no: chi ha governato dal 2001 al 2006 ha proseguito la politica di ripianamento delle perdite dell'Alitalia, con in più una leggerezza che voglio sottolineare, quella dei frequenti cambi di amministratori: in cinque anni, quattro consiglieri delegati e tre presidenti. Tra questi ultimi spicca il caso esemplare del presidente dell'Alitalia Bonomi, che, andandosene poi a Malpensa, non seppe fare di meglio che chiedere 1.250 milioni di euro di danni all'Alitalia per comportamenti lesivi messi in atto dalla stessa compagnia nei confronti di Malpensa, comportamenti ai quali evidentemente ha concorso egli stesso da presidente dell'Alitalia; vorrà dire che anche Bonomi dovrà pagare la sua quota di danni.

*articulo mortis*; proprio il Governo Berlusconi, nel luglio 2001, favoriva la stipula di un'alleanza tra Alitalia e Air France che, in vista di una futura integrazione delle compagnie, prevedeva uno scambio di partecipazioni, poi realmente effettuato l'anno successivo. Un mese prima dell'11 settembre 2001 l'Italia aveva visto giusto, aveva capito che l'Alitalia non poteva andare da sola ed aveva scelto come partner Air France. furono le incertezze del Governo ed i suoi dissidi interni a fare la frittata, quegli stessi dissidi di cui questa mattina i giornali danno conto all'interno del Governo della maggioranza.

Alitalia riuscì poco dopo a firmare un'intesa con Air France e KLM che nuovamente la proiettava sul mercato internazionale. È stata la nostra ultima occasione e venne sprecata anche questa. La condizione per rendere operativo il progetto era la privatizzazione di Alitalia, che non avvenne, come tutti sapete; niente privatizzazione, continua e progressiva perdita di quote di mercato e poi il vincolo europeo che ci impedì di ripianare le nuove perdite. Tralascio adesso di ricordare il danno che, sempre in quei cinque anni, per una dissennata politica che ha visto crescere in tutta Italia fino a 100 aeroporti, piccoli, medi e grandi, responsabili, tra l'altro, anche della crisi di Malpensa, come sapete. Oggi avrei voluto sentire questa verità

il senatore Legnini, l'ho confrontata con il ben diverso trattamento che il centrodestra riservò ingiustamente al dottor Angelo Rovati, per fatti che si sono dimostrati inesistenti e soltanto per colpire il suo rapporto con il presidente Prodi.

sostenuto da un azionista del settore dell'aeronautica civile capace di pilotare la compagnia fuori dalla crisi. Per noi questo azionista era Air France,

che il certificatore di Alitalia si appresta a non certificare il bilancio e che il nuovo presidente si appresta a dare le dimissioni, dunque è soltanto per senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori di Alitalia che noi voteremo a favore del decreto.

anche il Popolo della Libertà voterà a favore di questo decreto-legge, ma alcune osservazioni, anche in relazione agli interventi in dichiarazione di voto e in discussione generale - senza raccoglierne l'aspetto

che le sottoscriverei ancora. Mi ritrovo completamente in quelle dichiarazioni, credo che Alitalia sia una compagnia grande perché estremamente importante nel nostro Paese, ma piccola per competere nel panorama internazionale, quindi auspico che il all'interno di intese che ne rafforzino la competitività. Questa sarà una strada obbligata che il Governo dovrà percorrere se vorrà arrivare ad una conclusione positiva della vicenda. Al senatore Zanda,

voglio dire che è vero che negli anni del Governo Berlusconi abbiamo cambiato più volte amministratore delegato e che ci sono state delle

il sindacato e le aziende impostato in quel modo e quale fosse il ruolo del sindacato in ambiti così sensibili del pubblico servizio? però, che anche nei due anni del Governo Prodi sono stati cambiati tre amministratori delegati. Questa è una conseguenza delle difficoltà dell'azienda e forse oggi ripercorrerne

cioè dalla difficoltà del bacino di alimentazione degli aeroporti intercontinentali nel nostro Paese, e a questo veniva attribuito circa il 50 del valore delle perdite di Alitalia, cioè 150-200 milioni di euro. Non c'è dubbio che tutto questo avveniva anche perché il nostro sistema aereo non soltanto non aveva avuto la capacità di reggere nei confronti delle difficoltà a valle dell'11 settembre, ma non aveva avuto la capacità di adeguarsi al sistema *low che aveva cambiato radicalmente il sistema del trasporto aereo. Tutto ciò non è attribuibile all'Alitalia come azienda, ma è probabilmente un ritardo della politica a cui in questa legislatura siamo e saremo chiamati a dare delle risposte certe e rapide. Ricordo, tra l'altro, che sotto questo profilo esisteva un disegno di legge di riordino del sistema del trasporto aereo - tra l'altro presentato dal centrosinistra - che era dormiente da più di un anno in Senato.

allora dobbiamo liberarla dai gravami di Stato - su questo ritengo che siamo tutti d'accordo - per poterla vedere competere sul piano internazionale anche attraverso alleanze con altre compagnie. Il secondo tema concerne un sistema di riordino del personale. Sappiamo dobbiamo limitarne gli effetti e anche in questo caso il Governo dovrà intervenire con gli aiuti tradizionali che si danno in questo settore.

che consumano molto di meno dei vecchi aeromobili che sono patrimonio di Alitalia, quindi l'aumento del carburante non aiuta l'economia

è concretizzato; intanto, non c'era tempo di organizzare un diverso piano industriale e verificare se a livello di mercato ci fosse la possibilità di reperire capitali. di una classica situazione in cui l'aiuto di Stato non c'entra nulla. La Commissione europea a mio avviso non potrà che prendere atto di una condizione che i legali in genere chiamano *ad impossibilia nemo tenetur*. Non c'erano condizioni diverse per garantire l'esistenza in vita di questa azienda. Non è un aiuto di Stato, come hanno spiegato benissimo il presidente Grillo e il senatore Vegas.

*bipartisan*, un'azione di Governo resasi necessaria per una contingenza specifica, del tutto estranea a situazioni similari che hanno interessato i cosiddetti aiuti di Stato